i ministri Pinotti e Gentiloni hanno deciso di mandare dei soldati in Lettonia.

un'informativa presso la Commissione difesa e già allora domandai al Segretario Generale se era il caso di continuare la politica di allargamento della NATO verso la Russia.

pochi minuti fa, nella riunione della Commissione difesa, che ha trattato altri temi, mi sono permesso, nelle varie ed eventuali, di sollecitare una discussione su questo tema. Devo dare atto al presidente della Commissione difesa Latorre, che non vedo in Assemblea in questo momento ma era qui nel palazzo, aver risposto pubblicamente a una sollecitazione che, nei giorni scorsi, a nome del nostro schieramento, avevo pubblicamente avanzato, dando disponibilità in tal senso. senso. La comunicazione incidentale che sarebbe stata data a luglio nell'ambito della descrizione multi galattica delle missioni italiane non risolve la questione. Oggi, dopo il vertice di Bratislava e quanto avvenuto, l'eventuale presenza di militari italiani in Lettonia non è vista come una normale operazione di avvicendamento nell'ambito NATO, ma è apparso, come un segnale che aggrava la tensione internazionale.

relative alla Prima guerra mondiale. Vorrei che non arrivassimo senza discussione alla Terza guerra mondiale. E lo dico sapendo che non si corre questo rischio o, almeno, lo spero. Noi chiediamo che ci sia un'immediata discussione. Lo abbiamo detto pubblicamente nei giorni scorsi

sulla porta di casa (a calpestare i calli) di una forza che in questo momento è globale ed è effettivamente sotto pressione per una serie infinita di motivi.

proposta cui siamo favorevoli, ma ci permetterà di dire che forse non è il momento per fare simili passi. È un momento in cui il Segretario Generale della NATO dipinge la Russia come una nuova minaccia mondiale, e anche su questo bisognerebbe chiamare alla propria responsabilità il Segretario Generale della NATO. È un momento in cui il Presidente degli Stati Uniti ha ordinato alla sua struttura di *intelligence* di operare un attacco cibernetico al sistema strutturale informatico russo e, dall'altra parte, vediamo reazioni che potremmo definire anche responsabili da parte della Federazione russa. È un momento in cui sempre noi, appartenendo all'Organizzazione del Patto Atlantico, abbiamo dovuto seguire nella destituzione dei dittatori del Nord Africa, pensando di stabilizzare un'area, e ci siamo trovati con tutto il Mediterraneo in fermento. In un momento come questo, in cui l'ultimo obiettivo americano è la destituzione dell'ultimo dittatore dell'area mediterranea, al-Assad, sapendo che le forze russe, assieme alle forze governative siriane, sono ora le uniche che riescono a contrastare il pericolo globale, cioè il terrorismo internazionale: ebbene, pensiamo che, operando in questa maniera, destabilizziamo un sistema ci mettiamo veramente in una condizione di difficoltà di relazioni diplomatiche bilaterali con la Federazione russa. Pertanto chiediamo, come hanno il Ministro degli affari esteri o addirittura il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa insieme vengano a relazionare in Aula, perché la situazione è più grave di quella che siamo riusciti con poche parole a manifestare.

da quanto risulta, su richiesta di alcuni componenti dell'opposizione, la 5ª Commissione si è riservata ancora qualche ora per esprimere il parere sul testo e sugli emendamenti del disegno oggi all'ordine del giorno, e tenendo conto anche del fatto che la settimana scorsa non siamo riusciti a votare le ratifiche internazionali, alcune delle quali mi sembrano di una certa urgenza, pongo all'Aula la richiesta di un'inversione

Siccome io invece sono fiducioso che la maggioranza metterà la fiducia anche su questo provvedimento, voglio consentire alla maggioranza stessa di sciogliere il nodo.

«Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»

il disegno di legge in esame reca la ratifica del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro. Come ricorderete, il Montenegro, Paese di circa 700.000 abitanti, stretto fra i Balcani occidentali e il Mediterraneo e aperto all'influenza europea, dopo la dissoluzione dello Stato jugoslavo è rimasto legato alla Serbia, anche per la prevalente e comune impronta ortodossa, nella cosiddetta Repubblica federale di Jugoslavia, attraversando in maniera dolorosa tutte le fasi della guerra. Divenuto indipendente nel 2006, il Paese balcanico, forte di un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti e delle prospettive di ulteriore sviluppo economico che sarebbero potute derivarne, si è quindi risolutamente avviato sulla via della integrazione europea e atlantica.

Ad oggi il Montenegro, come ha riconosciuto la Commissione europea nel suo Country Report del 2015, ha compiuto progressi significativi in numerosi capitoli negoziali, tra cui quelli relativi al sistema giudiziario e diritti fondamentali e alla giustizia, libertà e sicurezza, sebbene debba ancora essere perfezionato sul fronte della lotta al crimine organizzato e alla corruzione. Altrettanto significativo, per quanto segnato da controversie in sede domestica, è stato l'impegno di Podgorica in direzione dell'Alleanza atlantica, nel solco peraltro di quanto già deciso da altri Paesi dell'area balcanica come Slovenia, Croazia e Albania. Alla decisione del Montenegro di aderire al programma denominato Partenariato per la pace con la NATO, avanzata sin dal dicembre 2006, hanno fatto seguito l'avvio di esercitazioni militari congiunte nell'Adriatico, l'invito ufficiale ad aderire all'Organizzazione formulato nel dicembre 2015

Si precisa innanzitutto come il fondamento normativo del Protocollo sull'adesione del Montenegro vada rinvenuto nell'articolo 10 del Trattato NATO del 1949, in base al quale le parti possono, con accordo unanime, invitare ad accedere all'Alleanza ogni altro Stato europeo che sia nelle condizioni di favorire lo sviluppo dei principi del Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione dell'Atlantico settentrionale. Il documento internazionale oggetto della presente ratifica, che si compone di un preambolo e di tre articoli, si limita dunque a regolare tempi e modalità dell'adesione del Montenegro nell'Alleanza atlantica. L'articolo 1, in particolare, dispone che il Segretario Generale della NATO, in nome di tutte le parti, comunichi al Governo montenegrino un invito ad aderire al Trattato dell'Atlantico del Nord. Il successivo articolo 2 disciplina i termini per l'entrata in vigore del Protocollo, stabilendo che, una volta ricevute tutte le notifiche previste dalle parti del Trattato, sia il Governo degli Stati Uniti a informare le stesse parti della sua entrata in vigore. Da ultimo, l'articolo 3 dispone che il Governo degli Stati Uniti sia il depositario del Protocollo. La ratifica oggi al nostro esame ha pertanto a oggetto non l'adesione sostanziale del Montenegro alla NATO, ma semplicemente l'invito ad aderirvi. A seguito della ratifica unanime di tutti i membri dell'Alleanza, si potrà poi procedere all'invito formale da parte del Segretario Generale della NATO al Paese balcanico. dallo scorso maggio - ripeto: dallo scorso maggio - siede nell'Alleanza atlantica in qualità di osservatore e partecipa già ad alcune missioni internazionali, potrà pronunciarsi in via definitiva sull'invito, scegliendo se divenirne ufficialmente il ventinovesimo Stato membro. Si tratta evidentemente di un evento di grande rilievo geopolitico, in una fase peraltro molto delicata per la vita dei Balcani occidentali. La situazione - com'è noto - è tuttora molto delicata in Paesi come la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo, né va dimenticata la difficoltà dei rapporti fra la Croazia e la Serbia. In ogni caso, si ritiene che il processo di allargamento della NATO in quell'area possa offrire condizioni di maggiore sicurezza e stabilità per l'intera regione dei Balcani occidentali e per la stessa zona adriatica, consolidando il processo di integrazione di quelle realtà nelle organizzazioni europee. Si fa inoltre presente che l'adesione alla NATO ha fortemente interessato la stessa opinione pubblica montenegrina, soprattutto la componente di origine serba. L'adesione di Podgorica, peraltro, è un tema che ha ripercussioni anche sulla politica interna: l'obiettivo prioritario della politica estera del Governo del *premier* montenegrino Djukanovic, *leader* del Partito democratico dei socialisti (confermato come partito di maggioranza relativa del Paese nelle elezioni politiche dello scorso 16 ottobre, con oltre il 41 per cento dei consensi), è da anni quello del progressivo avvicinamento alle strutture europee ed euroatlantiche. A tal proposito si ricorda che lo scorso 17 giugno, dopo la firma del Protocollo di adesione, il Parlamento montenegrino ha votato a maggioranza una risoluzione a sostegno dell'adesione del Paese alla NATO, quale viene ribadito l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione euro-atlantica, considerato una priorità strategica, rassicurando gli altri Paesi *partner* sull'affidabilità del futuro alleato e invitando al dibattito democratico i partiti anti-NATO che, nella realtà montenegrina, occupano una parte del fronte antigovernativo. In ogni caso, l'auspicio è che il processo di allargamento della NATO all'area balcanica, avviato da anni, possa proseguire senza strappi e senza dover costituire un possibile e ulteriore elemento di incomprensione con Mosca, con cui viceversa è opportuno - a mio avviso - rafforzare un dialogo costruttivo ai fini del consolidamento di un quadro di sicurezza internazionale più certo e definito. Concludo, signora Presidente, ricordando che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 3 articoli, che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Sono esclusi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La ratifica del Protocollo non comporta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. *(Applausi

Il *premier* Djukanovic, incurante delle proteste di piazza, non ha voluto nella maniera più assoluta sottoporre la decisione a un *referendum* nazionale, dichiarandosi immediatamente disponibile ad accettare la proposta di ingresso.

vanno avanti da secoli. Non è un caso che vi sia stata un'accelerazione nei tempi dell'adesione del Montenegro, perché poi, a seguire, sarà il turno di due Paesi che hanno un peso ben più grave negli equilibri geopolitici internazionali (mi riferisco alla Georgia e, soprattutto, all'Ucraina). Allora io dico no, a nome

di un'alleanza nata con scopi difensivi e di mutuo accordo tra i partecipanti, bensì di un'alleanza che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha visto salire in maniera esponenziale le azioni di provocazione, a

nello sviluppo della situazione economica e politica internazionale attuale. Esse vengono gestite in maniera unilaterale soprattutto dal grande alleato statunitense che, con le buone o con le cattive (spesso e volentieri con entrambe), veicola le decisioni dei Paesi aderenti alla NATO e le adesioni, soprattutto spingendo in maniera subdola e spesso nascosta con l'appoggio alle cosiddette rivoluzioni colorate.

è il caso di uscire dalla NATO o di far uscire la NATO dal nostro Paese, cosa molto più complicata.

democratica, partecipata e dal basso, su questo progetto di adesione. Pertanto invito il Senato della Repubblica, per quanto possa essere stato riferito qui in maniera davvero molto aleatoria dal collega che ha esposto la relazione introduttiva, a dire un no già in questa fase. Dobbiamo dare un segnale chiaro: non è necessario, in questo momento, che vi siano nuovi ingressi, in un'Alleanza che ha sempre più uno scopo di offesa nei confronti delle frontiere orientali dell'Unione europea. Si parla infatti delle aree già citate

vuole mandare, accendendo la miccia dell'enorme polveriera che si trova ai confini tra Ucraina e Federazione russa, allora la risposta può essere una soltanto: «Io dico no!». Senatore Petrocelli, non ho inteso interrompere il suo intervento, ma devo richiamarla, se mi può ascoltare, per stigmatizzare la gravità

con cui l'Italia ha in essere trattati importanti di collaborazione, da vari punti di vista, non ultimo quello della lotta alla criminalità, con tutto ciò che tale lotta rappresenta, nei rapporti con il

votato infatti per il rinnovo delle rappresentanze parlamentari e ha vinto il presidente uscente Djukanovic con un'alleanza di partiti, quindi in maniera molto più ampia e rappresentativa,

che ha sempre bisogno del Governo degli Stati Uniti per essere bollinato, rispedito e notificato. Abbiamo cioè capito che la NATO è un po' una propaggine degli Stati Uniti che ha la capacità e la possibilità di governare la geopolitica per la prima volta nella storia entra nella NATO uno Stato appartenente all'ex Jugoslavia,

siamo lì da una decina d'anni a tamponare le questioni kosovare, quelle del Montenegro in Bosnia. Abbiamo cioè una serie di antenne

Noi però non ci sentiamo di bloccare le aspirazioni dei montenegrini: se vogliono entrare in questa grande comunità, ci sembra scorretto dire che non hanno requisiti o titoli per poterlo fare.

il Montenegro all'interno della NATO, cosa significa pestare i calli alla Federazione russa dal momento che non lo ha conosciuto e se in questo momento storico debba prevalere l'interesse economico a quello della tranquillità di tutta l'area.

delle grandi pressioni americane nella NATO tutta l'Europa si è piegata a emanare una serie di sanzioni che per la prima volta nella storia non sono servite a punire il sanzionato, ma a penalizzare i sanzionanti. Veramente di questo non riusciamo ancora oggi a capacitarci. La distensione del Mediterraneo innanzitutto è un problema italiano. Tutta la questione immigrazione, derivata dalla destabilizzazione del Nord Africa, la sta pagando, qualcuno l'Italia. Si continua a seguire una politica che - percepiamo - va a ricercare, più che una guerra fredda, veramente una tensione oltre il limite tra Stati Uniti d'America e Federazione russa, Federazione russa, con la quale abbiamo sempre avuto e manterremo sempre buoni rapporti; un *partner* economico strategico per la pacificazione di tutto il Continente. Dobbiamo chiederci se i principi della NATO siano ancora validi. Se i principi della NATO erano quelli di potenziare una serie di Paesi da una possibile aggressione, allora vediamo che questi Paesi, spinti dalla testa della NATO, dagli Stati Uniti d'America, cercano un'aggressione nei confronti della Russia, e il Segretario Generale che viene a Roma - che non è Oslo - a predicare ad una platea come fossimo tutti anti-russi ha sbagliato completamente registro. L'Italia deve chiedersi se in questo contesto valga la pena fare un'ulteriore provocazione

se l'Italia ha ancora interesse a rimanere in una NATO che sembra volerci trascinare sempre più in un baratro, dove tutti gli interessi economici che prevalgono sono Oltreoceano e tutti i danni vengono pagati dalla parte che sta a Est dell'Atlantico.

è sempre stata e sarà sempre favorevole alle ragioni della solidarietà atlantica e alla NATO. È per questo che ci siamo anche schierati in maniera favorevole all'allargamento dell'Alleanza. pur confermando questo orientamento, l'occasione della conferma della nostra posizione a favore di questa adesione vuole servire a sottolineare quello che sta avvenendo, e si ricollega a quanto dicevo poc'anzi. La NATO

Non sono Matusalemme, ma sono abbastanza grande per ricordare le manifestazioni contro la dislocazione dei missili della NATO (i Pershing e i Cruise) al grido di fuori l'Italia della NATO, fuori la NATO dall'Italia! Qualcuno fa ancora queste manifestazioni, forse quando in Sicilia si mettono degli

quindi, da questo punto di vista, la posizione atlantica del centrodestra è molto chiara. Ho voluto fare un intervento su questo tema ricordando che, passando dalla storia all'attualità, qualche anno fa Silvio Berlusconi, che spesso è stato contestato anche per la sua politica estera, che è stata saggia e lungimirante, a Pratica di Mare, a pochi metri da Roma, portò la NATO a sottoscrivere dei patti con la Federazione russa. Ebbene, credo che Berlusconi, che ancora oggi è un protagonista della vita politica, nonostante le ingiustizie e le amarezze che ha dovuto patire, anche da parte di questa Assemblea, anche in questa legislatura ma questa è un'altra storia - ha cercato di comportarsi da *leader* politico italiano, da *leader* politico autorevole, perché non c'è bisogno di portarsi Benigni al seguito alla Casa Bianca perché poi c'è il rischio che non si sappia chi è il comico una volta arrivati alla porta della Casa Bianca! La NATO è stata interpretata dall'Italia del centro-destra in una maniera positiva di dialogo e gli accordi di Pratica di Mare sono stati un momento altissimo della politica estera italiana,

invece che una forza di sicurezza, di democrazia e di libertà, un momento di divisione. Anche perché quello che si sta verificando ce lo dimostra, e ripeto qui ciò che ho detto prima. Si dice: ma a luglio il Governo ha detto la tal cosa. Ma oggi questa operazione militare in Lettonia sta diventando un motivo di tensione e di divisione nel mondo,

la NATO, allora, ma attenzione a non farne un uso improprio. Il nostro voto è a favore, ma non certo della politica di questo Governo, bensì della politica che noi abbiamo fatto e che Berlusconi ha guidato, facendo della NATO strumento di forza, di democrazia ma anche di dialogo.

all'interno dell'atlantismo italiano in passato si siano confrontate due tendenze:

anche nel corso della guerra fredda riteneva che la nostra politica estera avrebbe dovuto trovare un suo baricentro e un suo ruolo in una posizione

Queste due linee ci potrebbero portare a ricostruire l'intera storia dell'Italia repubblicana, dalle sue origini degasperiane fino

ci confrontiamo con un nemico principale, che è il terrorismo internazionale di ispirazione islamica. Ci troviamo di fronte a una posizione americana che tende a un isolazionismo che attraversa le famiglie politiche americane molto più di quanto le contrapposizioni durissime di questi giorni potrebbero far pensare. pensare. La Russia, da un lato, è uno dei nostri principali alleati nello scontro con il terrorismo e, dall'altro,

che i conflitti vanno gerarchizzati e che, in altri momenti, le democrazie occidentali, forti delle loro ragioni, sono riuscite ad essere alleate, proprio per questo principio, anche con dittatori sanguinari come Stalin.

altra cosa è non prendere atto dei grandi cambiamenti del mondo, non discuterli e non assumere posizioni ragionate su tutto ciò. Visto che ci troviamo in una fase della vita di questo Senato, per

provvedimento in esame, per ragioni né particolarmente ideologiche, né legate a ragioni antiche, ma per una preoccupazione invece molto seria di come questa decisione possa incidere in maniera negativa su rapporti già molto delicati in politica estera, in particolare con la Russia. Vorrei ricordare all'Assemblea che nello stesso Montenegro questo provvedimento ha determinato una discussione complessa e non certo unanime, con posizioni, anche tra le forze politiche democratiche di quel Paese, decisamente differenti, con dubbi ed elementi che probabilmente avrebbero necessitato, anche da parte degli altri Paesi, un approfondimento maggiore e qualche cautela in più;

in un clima già teso e in una condizione che già nel corso di quest'anno, a partire dalla vicenda ucraina, ha visto una tensione dei rapporti

sull'adesione del Montenegro, come si è visto dagli interventi che mi hanno preceduto, ha suscitato un dibattito

che nella sua foga ha detto una grande inesattezza, perché non è vero che il Montenegro nei Balcani è il primo Paese che aderisce alla NATO, perché abbiamo Paesi dei Balcani che hanno aderito alla NATO, come la Slovenia, la Croazia

il problema non va visto secondo le lenti di ingrandimento della polemica politica, ma con estrema serietà. Cari colleghi, Gasparri prima e Quagliariello adesso hanno posto una questione che è seria, perché siamo di fronte a un problema che non va liquidato con l'occhio al 5 dicembre o a questioni interne italiane, perché altrimenti non ne verremo mai a capo. Noi abbiamo il problema, come Paese aderente alla NATO, di ridefinire ruolo, identità e futuro di un'alleanza che è nel codice genetico dell'Italia e del suo Parlamento. Dobbiamo stare attenti nel fare questo dibattito perché se diamo l'idea di essere dei pentiti della NATO non diamo certo un contributo alla serietà del dibattito Se non avessimo aderito alla NATO, saremmo semplicemente stati incapaci di realizzare anche quel poco - o quel tanto a mio parere - che l'Unione europea ha realizzato in termini di progresso, di benessere e di pace in questi cinquant'anni. La scelta europeista e atlantica dell'Italia, da De Gasperi a tutti i Presidenti del Consiglio che si sono susseguiti, è nel nostro patrimonio genetico. Oggi abbiamo un problema

Pensiamo al ruolo assertivo della Russia che è possibile grazie al vuoto che si è creato nello stesso Mediterraneo; pensiamo alla necessità di contrastare il terrorismo che è una nostra esigenza prioritaria,

che lo jihadismo e il terrorismo insidiano Russia e Cina potenzialmente non meno di quanto insidiano noi.

che è stata una bella cosa quella che fece l'allora presidente del Consiglio Berlusconi che lavorò perché si ampliasse il rapporto tra la NATO e la Russia. Però, diciamo anche la verità, oggi se vogliamo guardare e fotografare la realtà, dobbiamo attribuire anche ai russi qualche responsabilità. Pensiamo al cinismo con cui si stanno bombardando uomini, donne, bambini e famiglie ad Aleppo Est, altrimenti perdiamo di vista la dimensione della realtà. Mi interessa cogliere le parole dell'onorevole Quagliariello. Vogliamo fare su questo un grande dibattito? Credo sia utile che il Parlamento si esprima perché finalmente l'Italia deve portare il suo contributo alla definizione di un quadro più certo di politica estera. Concludo dicendo che stamattina ho partecipato, insieme al senatore Mauro e

alla domanda se si ritiene fondamentale un'integrazione più forte in Europa, gli stessi cittadini esprimono un giudizio positivo. I cittadini, in questo, si dimostrano molto saggi perché da un lato dicono di bocciare l'Europa per com'è, perché non è in grado di risolvere e di rispondere ai grandi quesiti odierni come l'immigrazione e la ripartizione degli immigrati. D'altro canto, però, gli stessi cittadini capiscono che senza Europa

tenendo presente la grande latitanza e difficoltà dell'Europa di oggi. Onorevoli colleghi, di questa NATO e di questa Europa non possiamo essere solo critici o spettatori. Noi ne siamo a pieno titolo protagonisti. Il nostro compito è rispondere alle sfide mettendo sul tavolo le nostre proposte. In caso contrario perderemo un'occasione storica.

Grazie fatico, pur avendo ascoltato con attenzione il collega Casini, a immaginare la ratifica di questa adesione alla NATO come un momento di protagonismo da parte del nostro Paese e del nostro Parlamento. La questione è centrale e non si tratta semplicemente di fare un dibattito anacronistico tra atlantisti e antiatlantisti. È evidente che l'Alleanza atlantica ha cambiato di segno la sua missione e non sempre si riesce a leggere come un'alleanza difensiva.

degli scenari in cui questi attriti si sono sviluppati, che non sono soltanto le recenti manovre in Lituania: il problema principale è come dobbiamo regolarci nel rapporto con la Federazione russa, anche relativamente alla più complessa vicenda che si sta dipanando in Siria e nella lotta al terrorismo.

Dubito che i contingenti del Montenegro possano arricchire la capacità persuasiva e deterrente dell'alleanza militare. Credo che si tratti, con tutta evidenza, di una decisione politica, che cade in un preciso momento politico e che rischia di acuire una ben definita e determinata tensione politica che sta attraversando il nostro sistema di relazioni internazionali. Credo che si debba segnalare un disagio. Signora Presidente, onestamente non ho mai creduto che si potesse essere atlantisti o antiatlantisti come si è di una squadra di calcio a un *derby*: della Roma o della Lazio.

di un sistema di alleanze che ha svolto la sua funzione storica, ma oggi siamo in un momento storico diverso e - vivaddio! - abbiamo la possibilità di concorrere, approfondendo tutte le questioni, affinché questo nuovo corso ci veda, non dico protagonisti, ma almeno coprotagonisti nel decidere chi siano gli amici e i nemici del momento di fronte alla sfida del terrorismo. Non credo sia stata un'enfatizzazione ricordare lo spirito di Pratica di Mare. La chiave delle relazioni internazionali, che ci può portare ad approdare a una una risposta più corale alle grandi sfide che vengono in questo momento dal grande arco di crisi, che va oramai purtroppo dalla Turchia fino alla Libia, passa attraverso quello spirito. Mi sento, quindi, nella condizione di dover sottolineare questo disagio ed è per questo che, in dissenso dal mio Gruppo, su questo provvedimento esprimerò un voto di astensione.

stata inutilmente compressa dalle acrobazie di calendario alle quali la maggioranza ci ha costretto già da una settimana e sia, quindi, in qualche modo casuale. È dalla scorsa settimana, infatti, che, per esigenze di coesione interna alla maggioranza, il nostro calendario sembra appeso al filo degli argomenti più inoffensivi tra quelli inoffensivi e la casualità, connessa alla bellezza e alla vivacità del regime parlamentare, ci propone la materia più inoffensiva tra le inoffensive, i trattati, con all'ordine del giorno la richiesta di discussione tra ambiti e limiti dell'atlantismo che si era affacciata in Assemblea già nella settimana scorsa. Non penso che il nostro Gruppo si possa sottrarre a questo, perché la memoria Grazie evocata da Casini, da Gasparri e adesso, con maggiore intensità, da Augello, l'abbiamo anche noi e l'abbiamo intatta. Però l'atlantismo è una cosa troppo grande, troppo diversa tra De Gasperi e Berlusconi, troppo diversa tra Pratica di Mare e oggi, di fare queste acrobazie sull'argomento Montenegro. Da questo punto di vista, io e il mio Gruppo voteremo a favore della proposta del relatore Pegorer. Lo facciamo con molta preoccupazione, perché non ci siamo distratti domenica, quando in Montenegro si è votato e ci sono state moltissime tensioni politiche, addirittura all'interno dei seggi. Fortunatamente c'erano attenti osservatori dell'Occidente (usiamo questo vecchio concetto, per me irrinunciabile per pensare la politica). Questo vuol dire che l'idea dell'adesione alla NATO è una speranza di stabilità e di stabilizzazione per quel Paese. Evidentemente le questioni della NATO sono molto più grandi e guardano a ben altro scenario che a quello balcanico, piccolo Montenegro o grande Serbia. Però non facciamo confusioni e sovrapposizioni di situazioni e di uomini. Ha ragione il presidente Casini nel ricordare come hanno guardato ad occidente Paesi che venivano dal comunismo nazionale di Tito. Però è questo il motivo per il quale, proprio ai tempi di Pratica di Mare, insieme a Gasparri, ad Augello e mi pare anche allo stesso Casini, eravamo molto critici circa la disinvoltura e la superficialità Grazie con molta disinvoltura e con molta leggerezza, senza approfondire niente di quell'idea originale di Europa che morì insieme alla morte fisica di Alcide de Gasperi e che era la Comunità europea di difesa, cioè l'Occidente democratico e antitotalitario per vocazione.

magari di destra, che sono più filoputiniani di quanto io sia stato filoamericano (e magari Casini con me); ma queste sono cose delle quali

sull'ordine dei lavori, vorrei apprezzare la discussione che avviene in quest'Assemblea, che andrebbe fatta molto più spesso. Purtroppo ci è permesso esclusivamente perché queste sono ratifiche: non contiamo nulla e quindi possiamo parlare. Assistiamo invece inermi alla Pinotti che vende armi

Sono presenti Benigni e Sorrentino: a qualcuno può piacere o non piacere il film «La vita è bella», che trattava dei campi di sterminio nazisti, ma certamente sono due vincitori di premio Oscar per i quali l'Italia dovrebbe provare un minimo di soddisfazione e di orgoglio.

Sulle questioni relative alle adesioni alla NATO ci sono state differenze e contrapposizioni profonde nell'Italia del dopoguerra. Se allora avessero adottato il criterio che qui molti hanno esposto, l'Italia non sarebbe entrata nella NATO, perché c'era una fortissima opposizione in Parlamento e nel Paese.

ci fosse un'unità rispetto ad alcuni valori, rispetto alla NATO, rispetto all'Occidente, rispetto a come stare nella NATO. Che ci sia bisogno di un dibattito generale e di fare il punto sull'argomento sono d'accordo, ma che si rischi di perdere per strada il cammino che è stato percorso e le conclusioni a cui siamo arrivati,

E tardi la comunità internazionale è intervenuta, perché anche in una comunità mondiale, come diceva Giovanni Paolo II, atti di ingerenza umanitaria o, come posso dire io, atti di polizia internazionale a volte sono necessari. Altrimenti si chiudono gli occhi e le orecchie di fronte alle stragi. Quel Parlamento e il Governo D'Alema si comportarono in coerenza con quanto decise la comunità internazionale. A chi non lo conosce chiederei, invece di fare battute, di leggere le riflessioni di una personalità come Alexander Langer. Che cosa diceva questo pacifista, cristiano e ambientalista rispetto alla questione della guerra nell'ex Jugoslavia? La pace non si può realizzare se non si guarda alla dignità, all'indipendenza e alla libertà dei popoli, perché se non si tiene conto di questi si ritorna al 1936-1938. Ci si illude, non guardando cosa succede, di realizzare la pace e invece si creano le condizioni per guerre che sono guerre distruttive. Il senatore Pegorer aveva già svolto una relazione - pensavo di fare un intervento breve quando ho ascoltato la sua relazione - in cui spiegava in modo concreto e chiaro cosa decidiamo oggi, qual è la decisione che prendiamo, il Protocollo d'intesa, le fasi previste nei tre articoli. Aveva sottolineato, come poi ha ripreso il senatore Casini, come ci siano

di fare questo percorso, noi diciamo no o diciamo sì. Questa è la domanda. Con chi stiamo? Con pezzi di piazza che contestano la democrazia rappresentativa e che contestano quel Parlamento, o con chi ha preso decisioni e si assume la relativa responsabilità perché in democrazia si fa così soltanto così si può decidere? Penso che per questo si debba decidere di sì e rispondere positivamente. Il Montenegro ce lo chiede perché lega a questa scelta la sua autonomia di Paese e non l'inimicizia verso gli altri. Ve lo immaginate il Montenegro che fa paura alla Federazione russa? Il Montenegro lo chiede per la sua autonomia, per il suo percorso in Europa e per rafforzare la sua democrazia. Questi sono i motivi.

si fa standoci o dimostrandoci pentiti? Si fa oggi pentitismo? Il Parlamento italiano fa pentitismo rispetto alla sua presenza. Come la pensate sulla cooperazione con l'Unione europea e sul fatto che l'Unione europea si sappia dotare di proprie forze armate e di un coordinamento? A prescindere dalla NATO o in cooperazione con essa? Se si pensa a prescindere dalla NATO, altro che riduzione delle risorse per le spese militari: ciò vuol dire moltiplicarle all'ennesima

anche italiane, operanti in quel Paese. L'intesa si compone di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo e si ispira al modello di convenzione fiscale dell'OSCE. Essa trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi. L'Accordo definisce il concetto di residenza, di stabile organizzazione, di redditi immobiliari e di utili di impresa, accogliendo il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Sono quindi stabiliti i criteri impositivi con riferimento ai dividendi, agli interessi e ai canoni. Articoli specifici disciplinano il trattamento fiscale dei redditi da servizi professionali e da lavoro subordinato, i compensi per gli amministratori e la materia delle pensioni. Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che cioè limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cile nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Gli oneri sono valutati in 425.000 euro annui a decorrere dal 2017, compensati però dai vantaggi che ne deriveranno negli anni per gli operatori economici. Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle nostre imprese e, in conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

nel Paese straniero in cui ha lavorato e che poi, alle finanze italiane, tocchi successivamente tassare solo le plusvalenze reddituali che

Tra l'altro, stiamo parlando di rapporti con il Cile, una delle economie emergenti dell'America latina con cui l'Italia ha anche rapporti profondi. considerate sono l'IRPEF, l'IRPEG l'IRAP, mentre per quanto riguarda la parte cilena sono quelle sul reddito e la rendita. Vengono così determinati criteri di attribuzione delle imposte gravanti sulle imprese e il modo in cui ripartire la stessa tassazione.

riguarda la rettifica del confine di Stato nel tratto del torrente Barbucina fra i comuni di San Floriano del Collio (in provincia di Gorizia) e di Obĉina Brda (in Slovenia). La piccola modifica del confine si è resa necessaria dopo i lavori di regimentazione del torrente, effettuati di comune accordo da Italia e Slovenia fra il 1986 e il 1993. Per questo è necessaria una modifica della Convenzione bilaterale del 2007 che ha finora definito

a parte quando Napolitano durante la commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine accusò ripetutamente i partigiani sloveni, tacendo sulla responsabilità dei fascisti per gli eventi della Seconda guerra mondiale, scatenando una vera e propria tensione diplomatica poi rientrata. Il motivo della mia agitazione è legato invece alla modifica dei confini. Proprio a febbraio di quest'anno, il Governo francese, infatti, ha temporaneamente preso possesso di una parte di mare italiano, in esecuzione di un accordo bilaterale con l'Italia, che non è ancora passato all'esame della nostra Commissione. La cessione del tratto riguardava una zona pescosissima, che avrebbe penalizzato i pescatori italiani. I francesi, poi, hanno riconosciuto che l'Accordo doveva ancora essere ratificato e hanno desistito. Capirà dunque, signora Presidente, che la mia preoccupazione era giustificata. Poi, ho visto il Trattato e mi sono rasserenata. Nel caso specifico, come già detto dai colleghi, si tratta di adeguare il confine di Stato alle mutate condizioni morfologiche Grazie

Signora Presidente, è veramente interessante sentir parlare di confini, come si sta facendo in questa ratifica,

invece crediamo sia una forma di fuga dalla realtà. Parlare di confini, di frontiere è parlare anche delle sottili differenze tra sistemi normativi, di valori, di progetti, di identità culturali, che possono, sì, certamente coesistere ma devono coesistere nel pieno, reciproco rispetto di diversità e sovranità. Riteniamo invece che l'assenza delle differenze rifletta una forma di imposizione di un modello dominante, che alla fine è quello dei Paesi più potenti e forti. forti. Il Gruppo Lega Nord voterà a favore della ratifica di questo Accordo, sperando ci sia anche una sorta di risveglio, che riporti il nostro Paese nella storia, liberandolo dall'illusione di utopie che in realtà non sono condivise

nei rapporti, positivi, con la Repubblica di Slovenia, la cui positività è stata anche favorita dall'intervento del presidente Napolitano in quei territori (esattamente la sensazione contraria rispetto a quella espressa

trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti, limitatamente all'imposizione sui redditi. Gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Sono stabiliti i criteri i criteri impositivi con riferimento ai dividendi, agli interessi e ai canoni. In materia di pensioni, il testo prevede in linea generale la tassazione soltanto nello Stato di residenza. L'Accordo prevede il ricorso al metodo di imputazione ordinaria per evitare le doppie imposizioni. Gli oneri vengono valutati

Presidente, anche io farò una breve dichiarazione per dire che, come Gruppo AL-A, votiamo a favore di questo provvedimento, perché anche questo, come il precedente, va nella direzione di favorire l'interscambio con un Paese importante con cui l'Italia ha questo tipo di

Signora Presidente, l'Accordo impegna le parti a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione per assicurare il rispetto della legislazione doganale, accertare e reprimere le violazioni di tale normativa e rendere più trasparente l'interscambio commerciale. L'intesa si compone di un preambolo e di 23 articoli e individua nelle amministrazioni doganali delle due parti le autorità competenti per la sua applicazione. Gli articoli da 3 a 7 disciplinano lo scambio di informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali. Sono previste anche particolari forme di cooperazione, dirette, tra l'altro, a semplificare i controlli doganali, ma anche a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti. L'articolo 13 impegna ciascuna amministrazione doganale ad avviare indagini, su richiesta, su operazioni doganali in contrasto con la legislazione doganale dell'altra parte. Ulteriori articoli disciplinano l'uso e la tutela delle informazioni ricevute, le ipotesi di diniego dell'assistenza e l'istituzione di una commissione mista. Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore. La spesa prevista è di circa 19.000 euro annui, per spese di missione e per le riunioni della commissione mista. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala, secondo la Commissione, criticità di ordine costituzionale, né motivi di incompatibilità con le normative europee internazionali, cui il nostro Paese è vincolato. Di qui la proposta all'Assemblea di approvarlo.

Signora Presidente, l'Accordo migliora, almeno nelle intenzioni, il controllo dei rapporti commerciali tra i due Paesi. Il Movimento 5 Stelle annuncia il voto favorevole,

L'Accordo è composto da un preambolo e da 15 articoli e ricalca nei contenuti altre intese della stessa natura già sottoscritte con altri Paesi. individua gli organismi istituzionali competenti per la sua attuazione nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e nella Direzione di pubblica sicurezza per la Giordania. principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa sono, tra gli altri: terrorismo, traffico di sostanze stupefacenti, criminalità organizzata, immigrazione illegale e tratta di esseri umani, traffico illecito di armi. È inoltre previsto che la collaborazione si estenda anche alla ricerca di persone sospette

e che venga assicurata la tutela dei dati sensibili trasmessi nell'ambito dell'Accordo stesso. L'intesa disciplina altresì le condizioni che possono determinare il rifiuto della collaborazione e prevede che le eventuali controversie interpretative o applicative fra le parti vengano risolte per via diplomatica. Il disegno di legge consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, autorizza una spesa complessiva di circa 160.000 euro annui. Il testo, a giudizio della Commissione, non presenta criticità di ordine costituzionale, né incompatibilità con la legislazione europea e con il diritto internazionale, e tiene conto delle disposizioni contenute in altre Convenzioni: tra queste la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e Convenzione ONU sulla lotta contro la criminalità organizzata del 2000. Sono queste le ragioni per le quali la Commissione propone all'Aula l'approvazione del testo.

aprile ho manifestato, a nome di tutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle, la nostra contrarietà all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Giordania, evidenziando come l'accordo prevedeva la cessione di navi, aeromobili, elicotteri, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine, razzi, missili e altro La Giordania è un crocevia per la fornitura di armi ai gruppi armati che combattono in Siria. Siamo certi che le armi che forniamo alla Giordania non vengano ceduti a terzi senza il nostro consenso? In attesa che si chiarisca meglio ciò che accade ai confini con la Siria, quello che il Movimento 5 Stelle intende per cooperazione tra Paesi è un'azione diretta ai fini della sicurezza e della pace. legge n. 2406, prevede invece la cooperazione tra le nostre forze di sicurezza e quelle giordane, che consiste principalmente in un costante scambio di informazioni tra le due parti. Da questo punto di vista, pur manifestando le nostre perplessità riguardo al ruolo della Giordania nello scacchiere mediorientale, non ci sentiamo di opporci a questa collaborazione auspicando che le nostre Forze dell'ordine e i nostri servizi di sicurezza sappiano gestire rapporti di questo tipo, rifiutando, ove ritengano, anche di fornire informazioni in conformità dell'articolo 14 del presente Trattato. Signora Presidente, io invece ritengo che questa sia una ratifica molto importante proprio perché la Giordania, oggi, in quello scacchiere e di fronte alla crisi siriana, rappresenta una Nazione di riferimento per cercare di stabilizzare

per cercare di essere incisiva nella lotta al terrorismo, nell'assistenza ai rifugiati e per quello che riguarda, appunto, la lotta alla criminalità. In questo, l'Accordo al nostro esame è molto positivo, quindi noi riteniamo che oggi debba essere approvato da quest'Assemblea. Grazie la materia è a noi molto cara ed anche delicata: parliamo della collaborazione tra forze di polizia. Ci rammarica il fatto che questo

com'è già stato detto, la Giordania è un Paese che riveste oggi un ruolo particolarmente delicato nello scacchiere mediorientale perché è molto esposto

ospita una quantità enorme di profughi. La collaborazione tra le nostre forze di polizia e le forze di sicurezza giordane è dunque un'azione per la pace in quello scacchiere. Il nostro voto, quindi, sarà convintamente favorevole.

*relatore*. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale. L'intesa, come altre già esaminate da questa Assemblea, è basata sostanzialmente sul modello modello predisposto dall'OCSE, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale e ha lo scopo di favorire la cooperazione fra i due Paesi attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale, necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. Composto di 14 articoli, l'Accordo costituisce tra l'altro il presupposto per potere inserire il Turkmenistan nella lista dei Paesi che consentono un adeguato grado di trasparenza fiscale. Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Non sono previsti oneri o minori entrate per le finanze pubbliche.

il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo del 2012 fra l'Italia e il Governo di Bermuda. Il testo segue il modello di intesa bilaterale di cui al precedente Accordo con il Turkmenistan. Il contenuto è sostanzialmente identico e quindi rinvierei alla relazione appena esposta, proponendo l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

tuttavia ci avvediamo che il provvedimento non è idoneo a superare l'ordinamento interno delle Bermuda, dove vi sono delle norme che consentono alle banche di non fornire informazioni sui loro correntisti. Per questa ragione,

fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005

L'estradizione è possibile per fatti punibili con una pena minima superiore ad un anno e per l'esecuzione di una condanna definitiva con una pena residua di almeno sei mesi. Com'è prassi internazionale, l'estradizione può essere negata per reati politici e per quelli che palesino nei confronti della persona richiesta un *fumus* di discriminazione. In nessun caso alla persona estradata potrà essere applicata la pena di morte. Viene inoltre stabilito il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona estradata non può essere perseguita, salvo alcune eccezioni, da parte dello Stato richiedente

e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale. Lo scambio di informazioni riguarda la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, è esatta percezione di diritti e tasse doganali

con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere così più efficace il contrasto alla criminalità. Di certo, l'intensificarsi dei rapporti fra l'Italia e il Cile comporta inevitabilmente che vi possano essere delle problematiche di natura giudiziaria e dei risvolti

Voglio solo cogliere l'occasione per precisare che nella precedente votazione sull'Atto 2468 tutto il Gruppo della Lega Nord si è astenuto.

da realizzarsi mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, nonché l'assistenza reciproca nella formazione del personale. Il testo disciplina altresì le attività di osservazione e inseguimento transfrontaliere, le consegne transfrontaliere, le forme di intervento comuni e il distacco di esperti per la sicurezza. Il Titolo IV disciplina le attività di cooperazione nella zona di frontiera comune, prevedendo anche una collaborazione nelle attività di rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento nonché il ricorso a forme di intervento comuni (inclusi i pattugliamenti misti), per le attività di prevenzione e contrasto della migrazione illegale. Le norme del Titolo VI disciplinano, sotto diversi aspetti, lo *status* giuridico degli agenti impiegati nel territorio dell'altra Parte rispetto alla responsabilità penale e civile. Gli oneri complessivi sono quantificati in circa 126.000 euro annui. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità e tiene conto degli strumenti giuridici di collaborazione già esistenti in ambito internazionale, fra i quali le Convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e contro la criminalità organizzata transnazionale. In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

sempre pronti a parlare di populismo, di salvaguardia dell'Europa, di libera circolazione e di tanti altri bei principi, la contraddizione palese che l'Accordo crea sotto le mentite spoglie della dicitura di accordo di «cooperazione di polizia». Scusate colleghi, ma non avevamo abolito queste frontiere dell'Unione europea? La ratifica dell'Accordo avallerebbe un atteggiamento palesemente antieuropeista, in un momento politico in cui l'Austria vive una profonda fase di instabilità politica che potrebbe favorire posizioni xenofobe contrarie all'interesse italiano. L'Italia e l'Austria sottoscriverebbero questo accordo quando, in realtà, al confine tra i due Stati si sono registrate gravi violazioni del diritto ai danni dei migranti, dei richiedenti asilo e, indirettamente, dei cittadini italiani già da diversi mesi. violazioni di cui l'Austria è pienamente responsabile e, a nostro avviso, il Governo italiano non ha fatto pesare in maniera adeguata questi errori alla controparte. Nonostante l'Accordo presenti elementi di cooperazione comunemente rintracciabili in altri accordi di questa tipologia, non ci sono in questo momento quelle condizioni politiche che ci porterebbero senza esitazione a votare sì a un accordo di questo

aggiungendo che l'Unione europea deve fare di più, ma anche che l'Italia sta facendo quanto necessario a garantire la sicurezza. Un passo indietro che dobbiamo valorizzare, soprattutto dopo le polemiche che sono seguite alla costruzione di un muro al confine con il nostro Paese nei mesi scorsi. Credo che il miglior modo per supportare le posizioni espresse dal Cancelliere sia, dunque, quello di non ratificare l'Accordo in esame, almeno per il momento.

intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla migrazione illegale, ai reati economici, al riciclaggio e alla criminalità informatica. Per questi motivi, il Gruppo AL-A voterà a favore del

Bisogna combattere insieme il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata, il commercio illegale di armi e droga e, nel caso di specie, anche l'immigrazione clandestina.

frontiera. Riteniamo che vengono fatti questi trattati e poi vengono eretti dei muri, forse quei muri che l'Italia stessa doveva aver eretto per quanto riguarda il problema della immigrazione clandestina. Sottoscriviamo

Quindi, ci troviamo nella contraddittoria situazione per cui in Istria e in Dalmazia la nostra minoranza riesce a fatica a garantire un minimo di di toponomastica e di bilinguismo, in zone che sono state italiane per secoli - penso all'Istria e a Fiume - mentre in Italia la minoranza tedesca, che deve essere assolutamente tutelata e che ha diritto ad avere i suoi nomi, che la Repubblica democratica gli ha garantito dal 1945 in avanti, sta cancellando

Non comprendo bene che cosa abbia a che fare questo Accordo internazionale con il problema della toponomastica

sul traffico illecito di stupefacenti, contro la criminalità organizzata transnazionale e anche sul controllo delle immigrazioni forzate. Si tratta quindi di un Accordo che entra positivamente in una dinamica problematica, ma che in qualche modo contribuisce a tenere in piedi il dialogo e ad affrontare una problematica così complessa come quella che in questo momento noi (e in seconda battuta l'Austria) stiamo vivendo sulla situazione migratoria.

Attualmente, la protezione dei brevetti è assicurata, anche negli Stati membri dell'Unione europea, dalla normativa interna o internazionale, in particolare dalla Convenzione di Monaco del 1973. L'Ufficio europeo brevetti si limita a facilitare la fase di rilascio del brevetto europeo, ma non prevede una procedura per il mantenimento in vita del brevetto, né adeguati rimedi giurisdizionali. Lo scopo delle nuove norme europee, incluso l'Accordo oggi al nostro esame, è quello di creare un sistema completo di protezione sovranazionale dei brevetti, con un'efficacia giuridica unitaria in tutto il territorio dell'Unione europea. Come i colleghi ricorderanno, l'Italia aveva inizialmente scelto (come la Spagna) di non aderire al brevetto europeo a causa dell'esclusione della lingua La nostra posizione è cambiata nel 2015, anche a seguito di alcune risoluzioni parlamentari e in base a una valutazione complessiva dei benefici delle nuove norme. Peraltro, come vedremo tra breve, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe consentire il recupero di un ruolo per la lingua italiana. La parte prima dell'Accordo concerne disposizioni generali e istituzionali, istituisce il tribunale unificato e ne definisce lo *status* giuridico e la struttura. Viene previsto un tribunale di primo grado (con la divisione centrale a Parigi e sezioni a Monaco e Londra, quest'ultima ovviamente da allocare in altra città), una corte d'appello e una cancelleria. I successivi articoli dettano norme sui criteri e le procedure di nomina dei giudici e sul loro *status*. La parte seconda dell'Accordo è dedicata alle disposizioni finanziarie, mentre la parte terza disciplina l'organizzazione e gli aspetti procedurali del tribunale Mi soffermo un attimo sul regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale. L'Accordo prevede, salvo eccezioni, che nei procedimenti può essere utilizzata una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata (che attualmente hanno sede a Parigi, Londra e Monaco). La sezione londinese sarà ovviamente cancellata con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. In vista dell'individuazione di una nuova sede, l'Italia ha sicuramente le carte in regola per candidarsi ad ospitare una sezione distaccata e in questo caso le verrebbe riconosciuto un ruolo di rilievo. Il disegno di legge in esame introduce anche delle modifiche alla normativa interna in materia di proprietà intellettuale e industriale per adeguarla alle nuove regole europee. Viene in particolare modificato il decreto legislativo n. 168 del 2003, che istituisce sezioni specializzate presso tribunali e corti d'appello, escludendo dalla cognizione di tali sezioni le azioni cautelari e di merito di competenza esclusiva del tribunale unificato. L'impegno complessivo di spesa per il nostro Paese, al netto delle minori entrate derivanti per l'erario, è stimato in circa 650.000 euro annui nella fase iniziale per arrivare, a regime, nel 2024, a circa 400.000 euro annui.

Signora Presidente, il voto favorevole a questa ratifica è dovuto anche al fatto che l'Italia, che è un Paese a propensione innovativa, nonché il quarto Paese europeo per numero di brevetti presentati, è anche un Paese particolarmente caratterizzato, nella sua innovazione e nei suoi brevetti, dalla presenza diffusa di imprese piccole, poco tutelate sul piano internazionale e che possono riferirsi normalmente esclusivamente al brevetto interno al brevetto interno del Paese come forma di tutela sui mercati internazionali, ben sapendo che è una forma di tutela ormai debolissima, anche se riconosciuta dalla Convenzione di Monaco del 1973. Il fatto che si metta in moto un meccanismo di riconoscimento europeo dei brevetti, pur con le difficoltà legate alla lingua che venivano sottolineate nella relazione - nei brevetti e soprattutto nelle parti descrittive e tecniche

a un percorso di valutazione di merito e giuridica europea uguale per tutti i Paesi. Quindi, proprio a tutela delle nostre piccole imprese, dichiaro

l'Accordo in esame ricalca il modello predisposto dall'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale e appare in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale. L'intesa, come altre già esaminate dall'Assemblea, ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale

i patrimoni di chi vuole evadere. Noi speriamo che ci sia un beneficio in termini di recupero di questa base imponibile sfuggita, anche alla luce della

fiscale e l'equità dei prelievi, cose che, purtroppo, nel nostro Paese non esistono più. In ogni caso, siamo favorevoli allo scambio di informazioni per rendere l'evasione sempre più difficile.

in un ambito di cooperazione multinazionale molto importante, anche dal punto di vista delle politiche internazionali del nostre Paese.

onorevoli colleghi, il Teatro Stabile di Genova, fondato nel 1951, compie quest'anno sessantacinque anni di vita e ieri, il 17 ottobre, sono iniziati i festeggiamenti di questo importante compleanno. Uno dei teatri pubblici più gloriosi d'Italia che ha una lunga storia, durante la quale lo Stabile ha costantemente rappresentato uno dei momenti più alti, a livello nazionale e internazionale, della cultura elaborata a Genova. Ancora oggi, il raggio di influenza del teatro tocca mediamente tra le 250.000 e le 350.000 presenze per stagione. A questi numeri, all'impressionante serie di *tournée* realizzate in giro per l'Italia, bisogna poi aggiungere che negli anni il teatro ha portato all'estero 27 spettacoli, mettendo in scena 383 rappresentazioni in 58 città. In Italia, questi dati, sono secondi solo a quelli del Piccolo teatro di Milano. Accanto all'attività di teatro, esiste poi la scuola di recitazione del Teatro Stabile, recentemente dedicata a Mariangela Melato e diretta da Annalaura Messeri. Tra i grandi attori che hanno collaborato a lungo con il Teatro Stabile di Genova, vorrei ricordare, tra i tanti, Enrico Maria Salerno, Alberto Lionello, Valeria Valeri, Gastone Moschin, Lina Volonghi, la stessa Mariangela Melato. Oggi purtroppo i finanziamenti pubblici sono sempre più incerti, con il rischio di mettere in difficoltà una realtà culturale storica la cui attività dovrebbe essere invece salvaguardata e preservata. E, allora, mi auguro che i festeggiamenti per i sessantacinque anni del teatro, che si svolgono proprio in questi giorni, siano l'occasione per conservare la memoria del teatro italiano e del Teatro Stabile, ma anche un modo per riflettere sul futuro dell'arte e della cultura in Italia, affrontando le sfide culturali che un mondo in continua evoluzione sottopone a noi tutti.

dell'incredibile voto con il quale l'Italia si è astenuta su una mozione dell'UNESCO che incredibilmente - lo ripeto - riscrive la storia dell'umanità.

distanziandosi da altri Paesi europei e dagli Stati Uniti, ha permesso di entrare alla rappresentanza palestinese, che non era ancora riconosciuta. Non sfugge a nessuno che dichiarazioni di questo tipo legittimino

Del Ministro degli affari esteri? Dove e quando si è deciso che l'Italia doveva votare mozioni che condannano Israele a essere attaccata e vilipesa negando le radici storiche della sua esistenza e della sua legittimazione ad esistere? Questa cosa non è passata inosservata. Domani ci sarà un *sit-in* davanti all'UNESCO. Tutte le persone, che ricordano non a parole la condanna dell'Olocausto del popolo ebraico, si indignano oggi nel momento in cui si ricorda

Signora Presidente, circa settantotto anni fa, in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento, venivano approvate le leggi razziali: un'onta indelebile nella nostra storia, ma almeno allora si rispettarono le forme. Si consultò il Parlamento, sia pure un Parlamento quale poteva essere quello formato in un'epoca di dittatura. Ma qualcuno ebbe modo di esprimersi e qualcuno non votò. Certo, chi si astenne commise un atto di ignavia.

quali passavano Gesù e i suoi discepoli per salire al Tempio, che era un tempio ebraico e non una moschea. Potrà sorprendere il Governo italiano, ma si trattava di un tempio ebraico, anche perché l'Islam è stato fondato quasi esattamente seicento anni dopo. anni dopo. Quel tempio ebraico non era un tempio ebraico qualsiasi, ma il centro, allora come oggi, come da più di duemila anni, della vita, del sentimento e della cultura ebraica. Ebbene, il nostro Governo, su una mozione di questo genere, si è coraggiosamente astenuto. L'ignavia è peggio della malvagità; e non c'è neanche in questo caso il

Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Giovanardi: questo non è solo un atto simbolico, ma un incoraggiamento ai terroristi ai terroristi e a coloro che vogliono cancellare con la violenza, con le bombe e con il sangue lo Stato ebraico, che - lo ricordo - è uno Stato delle Nazioni Unite prima dell'Italia. L'Italia è entrata nelle Nazioni Unite un po' dopo, perché aveva qualcosa da farsi perdonare, quell'abisso che evidentemente il Governo vuole approfondire con questo voto, che è una vergogna assoluta.

Il Governo, con un atto di disprezzo per la verità, per la cultura, per la religione di tantissimi italiani e per il Parlamento, ha deciso di mettere sotto i piedi tutto questo astenendosi astenendosi su questa vergognosa mozione. Chiedo quindi che il Governo venga a riferire su quanto accaduto. Sappiamo che è allergico a riferire, perché sono due anni e mezzo che aspetto una spiegazione dal Governo sul perché, sempre in sede di Nazioni Unite, votò contro un documento a favore della famiglie. famiglie. Speriamo che questa volta faccia un'eccezione, ma soprattutto che ci si penta ufficialmente - e davanti a tutti - di questo osceno e vergognoso voto che rinnova l'onta delle leggi razziali del 1938.